colleghi, la Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mattina, ha approvato modifiche e integrazioni al calendario corrente ed il nuovo calendario dei lavori fino al 28 ottobre. Oggi Oggi pomeriggio proseguirà la discussione della Decisione di finanza pubblica fino al voto finale. Ai Gruppi del Partito Democratico e dell'Italia dei Valori, che hanno esaurito i propri tempi, sono stati ulteriormente attribuiti 15 minuti ciascuno. Dopo il voto della risoluzione sulla Decisione di finanza pubblica, si passerà al seguito delle votazioni sugli emendamenti Dopo il voto della risoluzione sulla Decisione di finanza pubblica, si passerà al seguito delle votazioni sugli emendamenti al disegno di legge di riforma della professione forense.

Nella seduta pomeridiana di giovedì 21 ottobre, dopo l'informativa del sottosegretario Bertolaso sulle conseguenze dell'alluvione di Messina, avrà luogo lo svolgimento di interrogazioni. La prossima settimana, a partire dal pomeriggio di martedì 26 ottobre, il calendario prevede, oltre all'eventuale seguito della riforma della professione forense, la discussione di ratifiche di accordi internazionali e della mozione Pignedoli ed altri sulla politica agricola comunitaria e di eventuali altre mozioni connesse. Nella prossima riunione della Conferenza dei Capigruppo, da convocare nella giornata di martedì 26 ottobre, sarà definita la calendarizzazione della mozione Rutelli, D'Alia, Pistorio sulla politica economica, nonché nonché della mozione Li Gotti ed altri sul codice etico in tema di candidature elettorali.

accettata dal Governo, ed è iniziata la fase delle votazioni. Gli emendamenti già votati e quelli ancora da esaminare sono stati stampati e distribuiti. altresì che, prima della chiusura dell'ultima seduta, nell'esprimere il proprio parere sull'emendamento 5.3 e sui successivi 5.4 e 5.5, la relatrice si era rimessa al parere del rappresentante del Governo e quest'ultimo aveva invitato i firmatari al ritiro di tutte e tre le proposte emendative.

per una ragione strettamente attinente alla prosecuzione dei nostri lavori. A seguito della seduta di giovedì scorso, ho inviato una lettera al Presidente del Senato,

che dal Parlamento provengono al Governo a seguito di tale esame, ho scritto questa lettera al presidente Schifani, sottolineando tra l'altro che la vicenda che si era verificata poneva il Governo e il Parlamento di fronte ad una problematica giuridica ed istituzionale di assoluto rilievo, in quanto la legge di contabilità è chiara nell'affermare che, appunto, sono le risoluzioni parlamentari sulla decisione di finanza pubblica, e non il Consiglio dei ministri, a fissare i termini finanziari e gli obiettivi di saldo cui la legge di stabilità e la legge di bilancio devono attenersi. Proseguivo nella lettera dicendo che la deliberazione del Consiglio dei ministri mi appariva in questo senso adottata in spregio al ruolo che la legge di contabilità assegna al Parlamento, fino a prefigurare un evidente conflitto di attribuzione. Chiedevo al Presidente del Senato di adottare tutte le iniziative necessarie nei confronti del Governo per ripristinare il rispetto delle leggi che presiedono alle buone regole di finanza pubblica, materia peraltro costituzionalmente regolata, e perché venisse pienamente riaffermato il ruolo del Parlamento. Poi continuavo chiedendo che i provvedimenti relativi alla prossima manovra di finanza pubblica venissero approvati dal Consiglio dei ministri solo dopo l'approvazione da parte del Senato delle risoluzioni sulla Decisione di finanza pubblica. Ho avuto una prima risposta dal presidente Schifani con una cortesissima lettera arrivata a stretto giro nella quale mi si diceva che la mia lettera era stata trasmessa al Ministro per i rapporti con il Parlamento.

Voglio essere molto franca: non è questa la risposta che ci attendevamo dal Presidente del Senato. Non è la risposta che ci attendevamo perché la questione è radicata qui, dunque occorre che quest'Aula e il Presidente del Senato assumano una decisione che non appartiene in nessun modo e per nessun verso al Governo, né al Ministro per i rapporti con il Parlamento, né a quello dell'economia e delle finanze,

che il Senato abbia approvato la Decisione di finanza pubblica. La questione non può essere liquidata come un conflitto meramente politico, per una ragione essenziale, vale a dire che nel suo operare il Governo ha violato l'articolo 7 della legge n.

In questo senso è sintomatica l'apposizione del termine del 15 settembre per la presentazione alle Camere della Decisione di finanza pubblica, prima della presentazione, entro il 15 ottobre, alle Camere del disegno di legge di stabilità.

consultata dal Governo nel corso di questo procedimento, che pure riguarda la finanza pubblica. Peraltro, voglio ricordare che i lavori sono stati sospesi in quest'Aula giovedì perché la maggioranza per ben due volte ne ha avanzato richiesta. Vorrei

così come è stato affermato peraltro dalla Corte costituzionale con riguardo ai decreti-legge in base alla sentenza n. 161 del 1995, per affermare e preservare tempestivamente la competenza attribuita alle Camere.

Potrebbe opporsi, ma è un argomento del tutto non convincente, che il Governo ha violato una norma ordinaria, in questo caso l'articolo 7 della legge n. 196 del 2009. Però l'articolo 1, comma 4, della stessa legge fa un riferimento esplicito all'articolo 117 della Costituzione, una norma che si qualifica come principio fondamentale. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 27 del 1996, definendo la competenza costituzionale ha detto che essa può in concreto risultare dall'attuazione che le norme costituzionali abbiano trovato in norme primarie che con le prime facciano sistema. È chiaro

Il fatto poi che si tratti di un disegno di legge e di un atto non avente già forza di legge - mi riferisco al disegno di legge di stabilità - non è assolutamente dirimente poiché, ai sensi dell'articolo 37 della legge del 1953, istitutiva della Corte costituzionale, è ammesso ricorso persino in relazione a meri comportamenti, che valgono in quanto tali. Il costituzionalista Lucifredi ha scritto alcune righe molto interessanti in questo senso, affermando che l'istituto dei conflitti garantisce la consuetudine democratica, evitando la persistente invasione di un potere nella sfera di attribuzione degli altri e la formazione di quelle situazioni di predominio di fatto, che per lunga consuetudine diventano anche di diritto, che possono turbare l'equilibrio armonico dello Stato democratico aprendo la via alla dittatura. Detto questo, signor Presidente, credo ci siano tutte le condizioni,

per impegnare il Senato alla proposizione di un conflitto di attribuzione nei confronti del Governo. Altro che lasciare nelle mani del Ministro dell'economia o del Sottosegretario alla Presidenza la questione fondamentale che riguarda il ruolo, la funzione di controllo del Parlamento su una materia tanto delicata come quella della finanza pubblica, materia - lo ripeto - che trova nella Costituzione più di un rilievo e più di una regolamentazione oltre che una tutela.

Presidente, sottoscriveremo la mozione presentata dai colleghi del Partito Democratico. Mi permetto però di fare due considerazioni aggiuntive. La prima riguarda la seguente circostanza. Poiché la materia del bilancio dello Stato è riservata dalla Costituzione alla competenza del Parlamento, l'idea che ciò possa essere sottratto attraverso l'elusione della nuova legge che regola

il disegno di legge di stabilità prima che il Senato si pronunci sulla Decisione di finanza pubblica (cioè sull'atto di indirizzo generale cui il Governo si deve uniformare nella stesura della legge di stabilità) adducendo che deve rispettare il termine, è singolare, ridicolo ed offensivo nei confronti

e poi affermare che presenta la legge di stabilità il 15 ottobre per rispettare il termine, comprimendo il tempo assegnato al Parlamento per decidere sugli indirizzi di politica economica e finanziaria del Paese. Questo è vergognoso. Allora, anche dal punto di vista politico, abbiamo chiesto che il Parlamento sia messo nelle condizioni di svolgere una discussione vera sulle questioni economiche, anche alla luce di quanto sta avvenendo in Europa in questi giorni. Abbiamo quindi chiesto di inserire in calendario la mozione di cui è primo firmatario il collega Rutelli. Ma se ciò non avverrà, alla prossima riunione dei Capigruppo voteremo contro ogni calendario, da qui fino alla fine dell'anno. Non intendiamo, infatti, accedere alla tesi che la discussione pubblica sul bilancio dello Stato e sulla politica economica e finanziaria del Paese si faccia nei *talk show* e non in Parlamento. poi la circostanza che siamo in presenza non solo di una legge ordinaria, ma di una legge che dà attuazione ad un principio cardine della nostra Costituzione, il quale assegna al Parlamento il compito di approvare e redigere il bilancio dello Stato. Si tratta di un atto gravissimo di un atto gravissimo che nasconde l'incapacità politica di questo Governo di dirci cosa vuole fare in materia di politica economica e finanziaria e che non può passare sotto silenzio.

che non è in grado di approvare la risoluzione sulla Decisione di finanza pubblica. Immaginiamo, però, che questo stesso Governo, che non ha una maggioranza in Senato per approvare la Decisione di finanza pubblica tramite la risoluzione prevista dal Regolamento e dalla legge di contabilità, abbia invece la maggioranza per ottenere che l'Aula del Senato voti a favore di una sospensione dei lavori, modificando l'ordine del giorno dell'Aula, sulla Decisione di finanza pubblica. Quanto le sto descrivendo non è una ipotesi dell'irrealtà, perché è ampiamente possibile che accada.

‑ un emendamento, che nasce all'interno della sua maggioranza, che il Governo e il resto della maggioranza non vogliono approvare, ma non vogliono nemmeno disapprovare, perché altrimenti rischierebbero di non avere più la maggioranza sulla risoluzione complessiva sulla Decisione di finanza pubblica. Esiste però un orientamento della maggioranza, espresso dal relatore, favorevole alla sospensione dei lavori su quel punto. Ora, signor Presidente, lei che cosa direbbe se, utilizzando questa situazione che nasce da un deficit di rapporto tra Governo e Parlamento per quanto riguarda l'esistenza di una maggioranza necessaria per approvare la risoluzione sulla Decisione di finanza pubblica, il Governo approfittasse della decisione di sospensione dei lavori del Senato per approvare la legge di stabilità, la quale, in tanto può essere discussa e approvata dal Consiglio dei ministri, in quanto una risoluzione parlamentare, sulla base della legge di contabilità, contenga i limiti e gli obiettivi a cui la legge di stabilità e la legge di bilancio devono obbedire? Che cosa penseremmo noi del rispetto e della tutela dei poteri del Senato sulla decisione di bilancio nel suo rapporto con il Governo?

sulla legge di stabilità in assenza dell'atto di indirizzo - la risoluzione parlamentare sulla Decisione di finanza pubblica - che il Parlamento deve esprimere. Non è un'opinione, signor Presidente, ma è la lettura banale di ciò che prevede la legge di contabilità, la quale all'articolo 10, comma 1, stabilisce che «la Decisione di finanza pubblica, pubblica, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari, contiene gli obiettivi...» e così via. Di Di conseguenza non esiste una Decisione di finanza pubblica se non dopo la conseguente deliberazione parlamentare. Con il termine "parlamentare" si intende della Camera e del Senato, e non soltanto della Camera, ovviamente, almeno finché esiste il sistema bicamerale perfetto. che l'articolo 125-*bis* del Regolamento del Senato, al comma 4, prescrive tassativamente che il Governo, in Senato, al fine di evitare confusione,

Non è una questione di maggioranza e di opposizione, ma una questione di tutela del potere di decisione di bilancio in capo al Parlamento e, in questo caso, al Senato.

proviamo a sollecitare il Governo, la maggioranza e il Presidente del Senato affinché venga tutelato il potere di decidere sul bilancio da parte del Senato. non si tratta di una lotta tra Governo e opposizione, tra maggioranza e minoranza; la questione riguarda piuttosto la correttezza della procedura della decisione di bilancio, la madre (in termini di sede propria) dell'esistenza stessa di tutti i Parlamenti democratici che noi conosciamo. mozione. Il senatore Morando, invece, ha sollevato una questione di procedura proponendo sostanzialmente una questione sospensiva del dibattito in corso.

Signor Presidente, la presidente Finocchiaro, il senatore Morando e il presidente D'Alia hanno sollevato una questione

perfettamente argomentato la presidente Finocchiaro, che sarà calendarizzata nei modi e nelle forme previste dal Regolamento; altro conto è il problema che si è determinato, che è di enorme portata istituzionale, signor Presidente. Noi stiamo deliberando su una decisione che il Governo ha già assunto. Come dobbiamo comportarci? Il Presidente del Senato e il Governo prima che si apra la discussione e si voti su questo punto?

Quando è iniziata questa legislatura, il ministro Tremonti ha comunicato al Parlamento e al Paese che la stagione delle leggi finanziarie era finita.

Dopo questi nove minuti, che hanno preannunciato una rivoluzione nel rapporto tra Esecutivo e Parlamento e finalmente un meccanismo di stabilizzazione nell'esame, tanto più in pendenza della crisi economica e finanziaria globale, degli strumenti di politica economica e di bilancio da parte del Parlamento, che cosa è successo, signor Presidente?

Senza attendere che esso venga varato come prescrive la legge e nel corretto rapporto - non aggiungo una parola a quanto è già stato ricordato - tra Governo e Parlamento, il Governo ha varato la manovra per cui era obbligato a tener conto del parere delle Camere sull'ex DPEF. Ora ci troviamo in un punto nel quale, tra breve, il Governo porterà in Parlamento la manovra di bilancio,

fatto salvo il fatto che non siamo in condizione di fissare degli obiettivi strategici per la politica economica. Questo, come ricordava il senatore D'Alia, è l'oggetto di una mozione d'indirizzo legata alle politiche della crescita che un certo numero di parlamentari ha ritenuto di porre (e la condividerà) proprio per fare chiarezza in questo caotico processo che si voleva inteso a farla finita con le finanziarie *omnibus* e poi trasforma l'intero corso dei 12 mesi della vita del Parlamento in un *omnibus*. Questo è il tema. La richiesta di chiarimento al Governo su cosa intenda fare è pertanto ineludibile e credo sinceramente che seppure i colleghi abbiano desiderio, come ho fatto io, di dire la loro in questo passaggio così critico e al di fuori delle regole, ancora di più chiediamo al Governo di dirci dov'è il momento in cui il Parlamento assume le proprie determinazioni sulla politica economica, sul bilancio dello Stato, sui grandi indirizzi che riguardano la crescita. Questo è assolutamente decisivo, peraltro, da due punti di vista: alle decisioni che sono state prese nella notte da parte dei Ministri europei dell'economia e delle finanze relativamente al reindirizzo del Patto di stabilità e crescita europeo e quanto all'impegno, che ci coinvolge direttamente, che l'Europa ha definito

si deve pronunciare il Paese, si deve pronunciare il Parlamento. Non vi è traccia della strategia nazionale per la crescita che l'Italia deve configurare dentro l'obiettivo della crescita europea al 2020, strumento indispensabile perché il problema dell'Europa è la crescita. è la crescita. Dove sono le misure? Dove sono gli indirizzi? Dove sono le politiche? Ecco ciò che rende ancora più paradossale, signor Presidente, l'esame da parte del Senato di una litania di provvedimenti, ciascuno inconcludente e fine a se stesso, perché rinvia al successivo, ma nessuno dei quali rinvia al tema cruciale che tocca la politica economica del Paese, che è la crescita, la competitività, il lavoro, la tutela delle piccole imprese e della famiglia, su cui, di rinvio in rinvio, il Parlamento non discute, e di cui il Parlamento e il Paese nulla sanno. Se è vero quello che si è detto a proposito del ministro Tremonti, che egli goda di generale considerazione perché non dilata la spesa, in realtà noi di Tremonti constatiamo l'immobilismo nel mancato taglio effettivo mirato alle riforme del perimetro dei costi delle amministrazioni dello Stato e delle Regioni,

essendo io un parlamentare che ha votato la riforma dell'università. Noi votammo in quest'Aula la riforma dell'università sulla base del preciso impegno che vi sarebbero state le riforme, ma che vi sarebbero state anche le risorse. Senza risorse non ci sono riforme. Ci sono solo tagli lineari, si tradiscono gli impegni assunti davanti al Paese, si passa da un appuntamento all'altro e cresce la depressione e la sfiducia tra gli italiani. Questa è la materia del contendere. Non è un fatto procedurale, ma è la gravità della crisi economica che non vede risposte credibili da parte del Governo Signor Presidente, io non prenderò in esame l'ultima questione posta dal presidente Rutelli, perché attiene alla necessità di discutere nel Parlamento le nuove iniziative e la nuova regolamentazione della sessione di bilancio da parte delle autorità europee. È un problema senza dubbio di grandissimo rilievo

è necessario sia valutato poi dal Parlamento italiano e, quindi, nel nostro caso, dall'Assemblea del Senato della Repubblica. È una questione di rilevanza politica generale, sulla quale, ovviamente, si pronunceranno i Gruppi parlamentari, il Governo, la Conferenza dei Capigruppo e la Presidenza del Senato. Al contrario, interverrò sulle questioni poste dalla presidente Finocchiaro e dal senatore Morando che, seppur proceduralmente

della risoluzione sul documento recante la Decisione di finanza pubblica e, in particolare, sull'elemento essenziale e costitutivo, che sono i saldi ivi contenuti e che costituiscono, per il Governo, il limite entro il quale muoversi con la legge di stabilità e, per il Parlamento, i limiti alla emendabilità? Questa è la questione posta, e a questa io ritengo si debba dare una risposta. È ovvio che la strada maestra rimane quella della previa approvazione, da parte di entrambe le Assemblee, della risoluzione risoluzione con i saldi. Nella situazione contingente, però, si è verificato che, ad oggi, il Senato non ha ancora approvato la deliberazione. Voglio però osservare preliminarmente che la Camera ha già approvato la deliberazione e che i saldi previsti nella risoluzione del Senato sono identici a quelli della Camera. La proposta di risoluzione di maggioranza è stata presentata prima che il Governo avesse approvato la legge di stabilità, quando, dunque, era pienamente a conoscenza del fatto che entrambe le Camere proponevano, per l'approvazione, gli stessi identici saldi. Quindi, il Governo sapeva perfettamente questo, alla data del 15 ottobre, data stabilita dalla legge di contabilità perché il Governo approvi la legge di stabilità. Onorevoli senatori, voglio ricordare a tutti che esiste una fase parlamentare della nostra autonomia di assoluta rilevanza. Lo sanno bene i colleghi che, nel momento in cui dal Governo viene presentato - quest'anno alla Camera, a causa della turnazione, ma avrebbe potuto essere al Senato - il disegno di legge di stabilità finanziaria, esiste

La Camera dei deputati ha posposto, prima dell'assegnazione, questa fase, che, ricordo, viene pronunciata pronunciata dalla Presidenza del Senato sentita la Commissione bilancio, esattamente perché il processo parlamentare si concluda oggi con l'approvazione da parte del Senato della risoluzione con gli identici saldi. Sappiamo bene che è prevista una sanzione molto incisiva in quella sede: ove mai il Presidente della Camera trovasse uno scostamento tra i saldi, ne pronuncia lo stralcio. Sarebbe, questo sì, il caso in cui si troverebbe una difformità tra ciò che presenta il Governo e ciò che ha fissato la Camera. Invece, quando la Camera pronuncerà

dà inizio alla sessione di bilancio, che non a caso non è ancora cominciata. A me pare cioè che in punto di procedura - perché così è stata così è stata impostata la questione dalla presidente Finocchiaro e dal senatore Morando - sia una risposta una risposta assolutamente convincente quello che mi sono permesso in questo momento di sottolineare. È chiaro che è di gran lunga meglio se la si approva prima, ma credo questo è il punto specifico - che l'autonomia e la sovranità del Parlamento sulla decisione di bilancio non vengano assolutamente lese nel momento in cui parliamo, né lo saranno perché la Camera comincerà la sessione dopo la verifica dei saldi e dopo la risoluzione del Senato. Per concludere, signor Presidente, voglio dire che, sul punto, il Regolamento del Senato è identico a quello della Camera, nel senso che è prevista quella fase specifica e preliminare di verifica sul contenuto proprio anche al Senato. Questo, per chiudere il cerchio della corretta visione della situazione. Per questo, a me pare che si possano tranquillamente respingere le obiezioni proposte, con rilevanti argomenti, da parte dei colleghi della opposizione e che pertanto si possa votare contro la questione sospensiva richiesta dal senatore Morando. *(LNP)*. Signor Presidente, aggiungiamo qualche considerazione alle puntuali osservazioni del presidente Azzollini in merito alla procedura, consapevoli, certo, di trovarci in una situazione a dir poco anomala. Le nostre sono considerazioni di sostanza, ben ben sapendo che la forma ha comunque una sua rilevanza. Ebbene, il punto chiave è proprio quello dei saldi. I saldi, quelli sono e quelli rimangono. Quindi, avendo noi oggi all'approvazione una risoluzione sostanzialmente identica a quella della Camera - dove i saldi quelli sono e quelli rimangono - il punto chiave non viene viziato, a maggior ragione andando più nella sostanza del dibattito che ci interesserà da qui ai mesi successivi, avendo di fronte un documento finanziario elaborato dal Governo essenzialmente tabellare. Quindi, abbiamo come base di tabelle dei saldi. Cosa vuol dire tutto questo? Tutto bene? Certo che no. Noi siamo consapevoli che la situazione, per come si è evoluta, non è delle migliori. assolutamente e opportunamente la Conferenza dei Capigruppo ha all'unanimità proceduto verso il completamento dell'*iter* dell'approvazione della DFP e non poteva essere diversamente.

Poteva il Governo non procedere all'approvazione della legge finanziaria violando esso stesso la legge, perché poi c'erano dei termini da rispettare? Certo che no. Poteva il Governo non procedere all'approvazione della finanziaria per aspettare il Senato, rischiando di avere turbolenze sui mercati finanziari, cosa di cui sicuramente oggi non abbiamo bisogno? Certo che no.

Sarebbe stato sufficiente autoridursi i tempi delle dichiarazioni di voto e completare l'*iter* giovedì: così facendo, sicuramente avremmo reso un servizio al Paese e anche all'istituzione Senato che - come è stato fatto giustamente una sua rilevanza, un suo peso; e il Parlamento serve per decidere essenzialmente i numeri. Purtroppo non è andata così. Però, vediamola in positivo: abbiamo l'occasione di rimediare molto bene, proprio per come è attualmente organizzata la sessione di bilancio in relazione alla nuova sessione di bilancio europea, dove andiamo ad approvare una finanziaria che è puramente tabellare, dove di fatto abbiamo già discusso perché, come è scritto nella DFP, la finanziaria l'abbiamo già fatta a giugno. Il tema vero, tutto politico e di sostanza, è di lavorare insieme, magari con un po' più di buon senso di giovedì, nell'interesse del Paese per redigere un secondo documento. Quest'ultimo deve contenere il programma di riforme, indicando cioè come dare competitività al nostro sistema Paese, dato che i numeri quelli sono e quelli rimangono, e il nostro problema è recuperare ulteriori risorse e competitività per il sistema Paese. Abbiamo l'occasione di farlo

Presidente, replico molto brevemente alle osservazioni formulate dal presidente Azzollini, approfittando del tempo del mio Gruppo. Io spero che il presidente Azzollini, che stimo e con il quale ho un rapporto - mi permetto di dire - di amicizia, non si renda conto della gravità della propria affermazione nel momento in cui ha dichiarato: in fondo non importa che non sia intervenuta la deliberazione del Senato sulla Decisione di finanza pubblica, tanto la risoluzione di maggioranza recava gli stessi saldi. Mi chiedo, a questo punto, Presidente: noi qua che ci stiamo a fare? Glielo dico, perché mi pare che tutta questa discussione, questo ricorrere del termine procedura stia facendo sparire dall'orizzonte della nostra discussione la questione di cui stiamo parlando, e cioè che il Governo ha usurpato i poteri del Parlamento. È semplicemente questa la questione! Quindi, che cosa mi racconta che la risoluzione avrà gli stessi saldi? Peraltro, lei sa benissimo di essere omissivo: la Decisione di finanza pubblica e la legge di stabilità sono fatte solo di saldi, o per caso non sono fatte anche di misure qualitative qualitative - che sono le stesse sulle quali la maggioranza rischiava di spaccarsi giovedì scorso, sul Mezzogiorno, sui giovani, sulle imprese, sulle famiglie? Quindi, smettiamola con questa finzione: perché è una finzione. Il senatore Garavaglia è contento: beato lui! Chissà se sarebbero contenti i suoi elettori, senatore Garavaglia, nel momento in cui sapessero che questo Governo, nello scrivere e nel decidere la Decisione di finanza pubblica e la legge di stabilita, ha saltato a piè pari, mangiandolo, rosicchiandolo e divorandolo, l'articolo 117 della Costituzione (che per lei dovrebbe essere sacro) e ogni competenza, ogni controllo, ogni consultazione con le Regioni, le Province e i Comuni. Comuni. La questione è allora un'altra: qui c'è o no la necessità di sollevare un conflitto di attribuzione? Noi riteniamo che ce ne siano intere tutte le ragioni, e più vi arrampicate sugli specchi, più queste ragioni emergono solarmente. Dopodiché, permettetemi: se per caso le divisioni della vostra maggioranza conducessero ad un testo di risoluzione diverso, anche solo qualitativamente, da quello della Decisione di finanza pubblica, che si fa? Si ritira il disegno di legge di stabilità il disegno di legge di stabilità o si modifica in corso d'opera? Ma vi rendete conto che intervenire su un procedimento così delicato, sul quale - ha ragione il senatore Morando - sono nati i Parlamenti nell'Europa continentale, è un fatto di una gravità assoluta? Noi lo abbiamo evidenziato, con misura e con rispetto, invocando la presenza del Presidente del Senato, perché a lui spetta la responsabilità di difendere il ruolo e l'autorevolezza del Parlamento, maggioranza e opposizione comprese. senatrice Poli Bortone.

dall'identicità dei saldi, siccome il saldo è uguale alla Camera e al Senato, di conseguenza, secondo il presidente Azzollini,

un sillogismo un po' monco, perché la volta scorsa ci siamo accorti che quando finalmente il parlamentare assume tutte le sue prerogative, e quindi si sente libero dal vincolo di mandato, riesce persino a leggere un emendamento, a comprenderne il senso, a individuare un obiettivo e a sentirsi libero di votare per quell'obiettivo, che in teoria piace a tutti ma che, nella pratica, viene regolarmente disatteso. in mano un comunicato ufficiale della Presidenza del Consiglio che è stato diffuso esattamente un'ora dopo la sospensione della seduta della scorsa settimana. In quel comunicato, la Presidenza del Consiglio dei ministri fa sapere che il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge di stabilità per il triennio 2011‑2013 e il disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per il medesimo triennio e che tali provvedimenti, in linea

Ha anche la bontà di ricordare, laddove non l'avessimo ancora compreso (ora lo afferma proprio la Presidenza del Consiglio dei ministri), che la manovra economica finanziaria per il predetto triennio è stata in gran parte realizzata con il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Il che significa

sono più dotati di me di questo tipo di conoscenze, ma attingo al mio piccolo interessamento per questi argomenti),

che non c'erano e non potevano esserci, ma semplicemente per indicare degli indirizzi, pur se molto larghi ed a volte molto vaghi, in una procedura di decisione. Chi è stato parlamentare europeo peraltro sa qualcosina in Europa si fa (non è che non si faccia proprio niente): qualche strategia l'Europa la disegna, e nel disegnarla la indica ai Parlamenti. Tanto è vero che il nostro Ministro dell'economia ieri era molto contento di questo nuovo discorso

Non è solo quello: quelli sono obiettivi particolarmente importanti, ma l'obiettivo più importante qual è? È il tema della democrazia reale, che, in tanto si raggiunge e si verifica, in quanto c'è un rapporto corretto fra

che debbono convergere per creare una politica e dare delle linee convergenti di indirizzo. Non dobbiamo indicare delle cifre. Le cifre le fornirà il Governo, che si assumerà la

perché credo che il luogo della discussione non possa che essere questo. Anch'io mi appello al Presidente del Senato, il quale ha il dovere di tutelare la dignità

ma il dovere di intervenire per dare delle indicazioni. Stiamo chiedendo semplicemente questo. Perché se dovesse passare, ancora una volta, il *modus operandi* in virtù del quale si arriva in Commissione e si trova

ha introdotto un tema fondamentale che riguarda il ruolo e la centralità del Parlamento, individuando peraltro anche lo strumento attraverso il quale il Parlamento - in questo caso il Senato della Repubblica

qual è il ruolo del Parlamento nel suo rapporto istituzionale con il Governo su un tema così specifico e importante - il senatore

abbiamo bisogno di sapere come il Presidente del Senato è orientato rispetto ad una questione che riguarda il Senato.

che non sia nell'interesse di tutti condizionare i lavori del Senato ad un ragionamento di questo tipo, che potrebbe essere invocato tante altre volte creando soltanto la disfunzione di un organo che tutti noi siamo interessati a far funzionare meglio rispetto alla sua "dinamica" - a volte a volte collaborativa; in questo caso, e lo condivido, competitiva - in riferimento al comportamento del Governo.

la situazione di oggi può portare anche a polemiche strumentali. Voglio far presente due aspetti. La settimana scorsa abbiamo interrotto l'approvazione di questo provvedimento perché le opposizioni

Il secondo aspetto, colleghi, e mi rivolgo soprattutto al senatore Zanda per la richiesta che ha avanzato alla presenza del presidente Schifani in Aula: credo che questa sia anche una mancanza di rispetto nei confronti del suo Presidente di Gruppo. *(Commenti

presidente Belisario,

Il Gruppo del Partito Democratico ha sollevato un problema reale: stiamo portando a conclusione un dibattito che possiamo definire

Signor Presidente,

È chiaro che nessuno si vuole sottrarre alla discussione su questo argomento e nessuno ha inteso, soprattutto perché vi sono delle scadenze, chiedere di non discutere questo punto all'ordine del giorno. La questione in realtà è un'altra,

dalle conseguenti deliberazioni parlamentari - dunque di Camera e Senato - contiene gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica per il triennio successivo. Si pertanto di un atto complesso, che presuppone una deliberazione, peraltro conforme, dei due rami del Parlamento, che è preliminare e pregiudiziale all'adozione del disegno di legge di stabilità presentato dal Governo: lo dice con chiarezza la legge, che

le misure qualitative e quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10, e dunque riferiti alla Decisione di finanza pubblica. Pertanto, se non si conosce qual è la Decisione di finanza pubblica deliberata conformemente da Camera e Senato, come si può esaminare la legge di stabilità? Ed ancora, riferendomi ai colleghi della Lega, grandi federalisti, poiché la legge di contabilità è stata predisposta anche per armonizzare i bilanci dello Stato con quelli delle Regioni e degli enti locali

che è stato presentato illegittimamente, in violazione di una procedura normata da legge ordinaria, ma di rilievo costituzionale per i suoi riflessi sugli articoli 81, 117 e 120 della Costituzione),

illegittimità della legge di stabilità che la Corte, qualora adita da un qualunque giudice, potrebbe rilevare. Io mi chiedo se convenga, per prepotenza, correre il rischio di dare vita ad una legge di stabilità, in un momento peraltro così difficile per il Paese, che reca in sé il germe della illegittimità. Detto questo, abbiamo richiesto la presenza del presidente Schifani, non soltanto perché non capita ogni giorno di discutere in merito ad un conflitto di attribuzione, ma anche per una ragione assai più precisa e di fatto. Innanzitutto, è stato il presidente Schifani - credo anche in assenza di un voto - che nella scorsa seduta ha dato il via libera al rinvio della discussione oltre il termine nel quale il Governo era tenuto, per legge, a presentare il disegno di legge di stabilità:

ha ritenuto di rispondere a questa nostra sottolineatura, che chiamava in causa la Presidenza e il Senato, dicendo di aver trasmesso la lettera al Ministro per i rapporti con il Parlamento.

Peraltro, voglio osservare che qualora approvassimo la Decisione di finanza pubblica *telle quelle*, ammesso che la maggioranza possa permetterselo - e immagino che in condizioni d'emergenza se lo permetterà - daremmo vita ad una decisione inutile e che non sana l'illegittimità. Non la sana retroattivamente, collega Azzollini, perché il punto non è se la deliberazione è uguale al disegno di legge di stabilità: il punto è che il Governo deve tenere conto dell'indirizzo del Parlamento. venisse modificata, mi chiedo che cosa farebbe. Il Governo: ritira il testo? Ne presenta un altro, o presenta emendamenti? Come sana questo *vulnus*? Si tratta di una questione delicata, anche perché è la prima volta in assoluto

Ovviamente ciascuna forza politica, il Parlamento e la maggioranza, si assumono le proprie responsabilità nelle decisioni che prendono. Noi abbiamo il compito

che, nel recente intervento sulla crisi, il Presidente del Consiglio si è solennemente impegnato a realizzare, a partire dalle infrastrutture e dalla fiscalità di vantaggio;». **(6-00041)

è impegnato non soltanto a fare ciò che ha detto quando gli avete concesso la fiducia, ma in particolare a dare priorità priorità al tema delle infrastrutture e della fiscalità di vantaggio. Si tratta di due temi ai quali teniamo moltissimo. La perequazione infrastrutturale per noi meridionali è un fatto di primaria importanza: non devo certo dirlo a lei, Presidente, che è meridionale come me e quindi sa perfettamente quanto sia importante che un terzo dell'Italia non venga emarginato, il che richiede che prima dell'applicazione del federalismo fiscale si intervenga realmente attraverso la perequazione infrastrutturale. Altrettanto importante è la fiscalità di vantaggio, che era stata promessa dal Governo ma rispetto alla quale, fino a questo momento, non abbiamo ancora avuto alcun segnale. Dunque, chiedo conferma ai colleghi, a partire dal presidente della

caso manteniamo il testo con questa formulazione e ritiriamo i due emendamenti sull'agricoltura, non perché si voglia agevolare oggi certi percorsi del Governo, ma semplicemente perché in Conferenza dei Capigruppo

del sistema agroalimentare e un intervento per i contributi agricoli unificati, in particolare per quanto attiene alle aziende agricole del Mezzogiorno d'Italia.

cambiamento delle parole «impegna il Governo» con le parole «a dare seguito» per me non muti la sostanza né dell'emendamento né dell'accordo. Pertanto, per quel che mi riguarda, ribadisco quanto ha dichiarato la senatrice Poli Bortone. Noi voteremo a favore di questa riformulazione dell'emendamento e la senatrice Poli Bortone ritirerà gli emendamenti successivi, così come concordato. Presidente, vorrei anticipare il nostro voto favorevole rispetto alla proposta emendativa della senatrice Poli Bortone,

di grande portata politica, che ci costringe a tornare sull'argomento che abbiamo appena finito di discutere.

contiene non solo le misure quantitative necessarie al conseguimento degli obiettivi programmatici, ma anche quelle qualitative, così come definite dalla Decisione di finanza pubblica integrata dalle risoluzioni parlamentari. Abbiamo appena integrato la risoluzione parlamentare approvata dalla Camera con un emendamento che contiene misure qualitative, in termini di indirizzo, di portata enorme, perché si tratta della fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno, che il Governo è impegnato a contenere dentro la legge di stabilità, e delle misure relative alla costruzione di nuove infrastrutture nel Mezzogiorno.

di forma, essere accettato. La norma, però, dice che la legge di stabilità deve contenere le misure qualitative necessarie per realizzare gli obiettivi programmatici fissati dalla risoluzione sulla Decisione di finanza pubblica; e noi abbiamo inserito nuove misure qualitative. Il problema è chiaro: la Decisione di finanza pubblica, così come esce dal Senato, è diversa su questo punto fondamentale da quella che è uscita dalla Camera, e la legge di stabilità, così come definita dal Consiglio dei ministri della scorsa settimana, non è corrispondente alla legge di contabilità viola apertamente lo stesso Regolamento del Senato, e ciò, non per quello che riguarda la procedura seguita dal Senato, che è corretta, ma per quanto riguarda il rapporto tra la decisione del Senato e la decisione del Governo, risultando chiaro che il Governo ha a questo punto *per tabulas*, essendo stato introdotto questo emendamento, violato palesemente nel loro nesso l'articolo 11 della legge di contabilità e l'articolo 125-*bis* del Regolamento del Senato, tra di loro connessi in modo indissolubile.

per chiedere al Presidente del Consiglio o al Ministro dell'economia di venire in Aula per annunciare il ritiro della legge di stabilità e, naturalmente, di riunire di conseguenza il Consiglio dei ministri per approvare una nuova legge di stabilità coerente con la decisione assunta dal Parlamento. *(Applausi dal

vorrei chiedere, se è lecito, alla relatrice e al Governo di darci un'indicazione su come procedere. Non ripeto le cose che sono state già dette dal senatore Morando, ma è evidente che ci troviamo di fronte ad un testo approvato dal Senato che modifica la Decisione di finanza pubblica così come sottoposta dal Governo alla Camera ed al Senato. Quindi c'è una deliberazione non conforme, non conforme, non univoca, tra Camera e Senato e c'è una legge di stabilità presentata in Parlamento sulla scorta della deliberazione della Camera, che non tiene conto della deliberazione del Senato. prima ancora che politico è di natura squisitamente procedurale, e spero e mi auguro che lei, con la sua sensibilità, ci aiuterà a scioglierlo: come procediamo dopo questo voto al Senato?

che ha modificato - in maniera positiva, dal nostro punto di vista - la Decisione di finanza pubblica, ma che è una deliberazione diversa da quella adottata dalla Camera, e a sua volta è una deliberazione diversa da quella propedeutica alla legge di stabilità già presentata alla Camera.

ma per comprendere quale fosse il percorso più efficace per mettere il Parlamento nelle condizioni di esprimere l'atto più importante dal punto di vista economico e finanziario che è la Decisione di finanza pubblica. Il Senato ha modificato la Decisione di finanza pubblica; lo ha fatto dopo che la Camera ha adottato un altro testo e dopo che il Governo, strafregandosene della deliberazione del Senato, ha presentato un testo conforme a quello della Camera. La domanda quindi è molto alla Camera per essere votata, si ritira il testo della legge di stabilità e lo si adegua a queste decisioni? Almeno su questo, credo che il Governo e la maggioranza una parola di chiarezza ce la debbano dare, e lo debbano fare ora, perché ci accingiamo a dare il voto definitivo su questo documento e non sappiamo qual è il suo valore, quale effetto e quale rilievo avrà nel procedimento. Ciò, anche alla luce del fatto che, come ho detto in precedenza, la Decisione di finanza pubblica condiziona i bilanci i bilanci delle Regioni e del sistema delle autonomie, perché è atto propedeutico non solo alla legge di stabilità, e quindi alla legge che governa il bilancio dello Stato, ma è atto propedeutico alla redazione e all'approvazione dei bilanci degli enti locali, i quali si trovano di fronte a due decisioni: una adottata dalla Camera e una adottata dal Senato. Quale delle due devono prendere per buona? A quale si devono uniformare? Oppure tirano i bussolotti e, a seconda che si trovino a Nord o a Sud, adottano l'una o l'altra come punto di riferimento per il bilancio? Almeno questo, siete capaci e in condizione di dircelo?

Adesso, si è arricchito di elementi sostanziali. Come ha spiegato bene il senatore Morando, il Parlamento, nella sua piena consapevolezza, aveva già avuto un passaggio anticipatorio la settimana scorsa, quando si è espresso

Il problema, obiettivamente, determina ora delle conseguenze per quanto concerne questo documento, vista la premessa così articolata relativamente al passaggio della settimana scorsa.

diffusa è un rito assolutamente incapace di produrre effetti sostanziali, e attorno a un rito incapace di produrre effetti sostanziali si possono anche concedere momenti rispetto a proposte di piccoli Gruppi o, addirittura, cercare una fase parlamentare condivisa. Non tocca a me svelare l'arcano e sciogliere il nodo tecnico e giuridico che si è determinato. Io voglio solo ribadire Sapendo che di vincolante in questa vicenda non vi è nulla; che il rapporto fra Parlamento e Governo è fortemente sbilanciato; che tutte le questioni, assolutamente pertinenti che sono state poste, troveranno una sede parlamentare con la mozione sul conflitto di attribuzione, io comunico solo che, per quanto riguarda me, il mio piccolo Gruppo, il mio movimento politico, il Movimento per le Autonomie, noi riteniamo il Governo vincolato politicamente a questo documento. Quanto ci interessa è che in Parlamento, a grande maggioranza, anzi all'unanimità, è stato detto al Governo che se vuole essere fedele agli impegni sanciti con gli elettori e affermare davvero un programma che abbia come obiettivo lo sviluppo del Mezzogiorno deve procedere con un grande piano infrastrutturale in adesione alla legge delega sul federalismo, che prevede la perequazione infrastrutturale (come ha detto benissimo la senatrice Poli Bortone) e deve avviare una seria fiscalità di vantaggio. Per me ciò che rileva questa sera è che nei rapporti di maggioranza, cari amici della Lega contano gli impegni sanciti in Parlamento. Troppe volte questi impegni sono stati violati: ora, siccome mi è stato riconosciuto di essere un po' leghista, io farò come i leghisti, pretendendo che l'impegno sia rispettato, come per il federalismo e come per altri impegni. Questo è quanto volevo dire, pur sapendo che su questo provvedimento noi non potremo far gran conto, malgrado esso sia stato definito con la massima solennità.

stamattina che sono stati definiti nuovi criteri molto più flessibili, che lasciano spazio all'intervento della politica evitando al nostro Paese una condizione di forte rigidità e la necessità di misure durissime sul tema della finanza pubblica, visto l'impegno di riportare il debito intorno al 60

che i risultati ad oggi sono insoddisfacenti: vi sono ad oggi la necessità di manovre correttive e non certamente di tipo solo tabellare

e concludo, che il documento in quanto tale ci lascia ampiamente insoddisfatti. Lo definiamo insoddisfacente, reticente, inadeguato e superato; però, lo riteniamo da stasera, con le dichiarazioni che ha reso il Presidente del Consiglio in Parlamento, alla Camera e al Senato, con cui si è impegnato sui cinque punti a svolgere un'azione di grande riforma (dal fisco fisco alla giustizia, ma anche sul Mezzogiorno), che possono consentire di liberare risorse e garantire una prospettiva di sviluppo. Ma l'impegno che il Parlamento ha indicato al Governo affinché inserisca nelle misure di finanza pubblica la fiscalità di vantaggio per il Sud ed un piano per le infrastrutture ci consente di votare questo provvedimento, che di per sé sarebbe del tutto insoddisfacente.

il senatore Morando poco fa ha proposto, a seguito di un fatto nuovo, molto importante, una nuova questione sospensiva e lei ha dato corso a quella discussione.

Perché il Senato decide nella sua totale autonomia; il Governo si assumerà le sue responsabilità. Noi intanto abbiamo preso una decisione. *(Commenti

lei non aveva e non si è pronunciato in modo chiaro e motivato su questa questione. E siccome non è una proposizione dilatoria, ripropositiva di argomenti già svolti, ma è stato detto, e ribadisco, che siamo in presenza di un fatto nuovo, senza precedenti, in quanto l'Aula del Senato poco fa ha approvato un emendamento che modifica la risoluzione di finanza pubblica, ed obbliga il Governo a modificare la legge di stabilità, quanto meno, signor Presidente,

per le ragioni che ha ricordato la presidente Finocchiaro prima. Ci vuole dire qualcosa il Governo? Si vuole alzare il Governo e dirci se ritira la legge di stabilità, non tiene conto di questo voto? Una cosa ce la deve dire. Ribadisco: siamo in presenza di una pagina eccezionale nella vita del Parlamento.

nel contenuto del suo intervento, nell'ambito di una procedura che riguarda le nostre decisioni, inserisce di continuo la richiesta che il Governo intervenga. Questo è un profilo che a noi come Senato non interessa.

Presidente, ci devono essere le condizioni per parlare, anche perché vorrei utilizzare il tempo disponibile

alcune linee importanti di politica economica e una visione di insieme, oltre all'esigenza di riforme strutturali per sciogliere il nodo della crescita); al senatore De Angelis (che ha sviluppato una riflessione attenta e ponderata sul federalismo e sul suo impatto finanziario, e ha segnalato l'importanza del recupero di protagonismo delle parti sociali e del ruolo che stanno svolgendo, per cercare di riportare

sviluppo e interveniamo su alcuni nodi fondamentali e importanti); a quanto segnalato dal senatore Valditara nel suo intervento in riferimento all'istruzione e all'università all'esigenza, che non può essere tralasciata, di accompagnare la riforma con le risorse necessarie per consentire che la stessa si concretizzi e risponda alle richieste che da più parti arrivano di far finalmente entrare in vigore la riforma dell'università) e dalla senatrice Germontani (che ha posto in particolare l'accento

della maggioranza stessa sulla centralità dello sviluppo del Mezzogiorno, a partire della questione infrastrutturale e dalla fiscalità compensativa,

peccato che l'opposizione si sia fermata alla questione fondamentale di carattere procedurale e non abbia deciso di accompagnare e condividere la questione politica positiva emersa dalla maggioranza ampliata con il concorso degli altri soggetti Governo, abbiamo assistito in queste ore ad un dibattito importante che pone al centro dell'attenzione la centralità del Parlamento.

inversione e perversione dei ruoli costituzionali, per cui non è più il Parlamento che controlla il Governo, ma è il Governo che controlla il Parlamento, ha scritto in il Parlamento, ha scritto in maniera molto chiara nella premessa della Decisione di finanza pubblica che il documento è sostanzialmente e politicamente superato.

Ci è stato inoltre detto che il documento avrebbe avuto una qualche attualità in occasione delle decisioni che si sarebbero assunte a livello europeo. consideriamo assolutamente credibile la soddisfazione che il ministro Tremonti ha espresso in seguito ai risultati dell'accordo quadro di ieri,

ieri. Infine, perché in questa ricerca di equilibrio tra il rigore dei conti pubblici e la crescita del Paese noi non riusciamo a vedere nessuna proposta seria e credibile. dire, quindi, che dal dibattito che si è svolto su questo documento inutile - come è stato ripetuto già ampiamente - emerge semplicemente la lenta ed inesorabile agonia politica di questa maggioranza. Questo è l'unico dato di fatto. Il capolinea a cui è arrivata a cui è arrivata questa maggioranza è fatto di chiacchiere, di caos e di rotture: rottura con la Banca d'Italia che, nell'evidenziare una situazione seria e non certo facile per il nostro Paese, viene accusata di dare numeri esoterici ed ansiogeni; rottura con la Confindustria, con chi sino a poco fa era il vostro interlocutore privilegiato e che ora denuncia ribrezzo e schifo per questa politica avvelenata ed inconcludente; rottura tra i Ministri, con la Gelmini che scopre di non avere risorse per realizzare la riforma dell'università, la Prestigiacomo che non vuole passare alla storia come il primo Ministro dell'ambiente che ha chiuso i parchi, e Bondi che è stanco di essere fischiato ovunque vada perché qualcuno gli ha detto che con la cultura non si mangia; rottura con le stesse tre gambe della maggioranza sulle grandi questioni, come la questione del Mezzogiorno, dove è bastata la proposta di un semplice correttivo ad una risoluzione priva di valore di vincolo di legge per far capire che l'unico piano per il Sud di cui questo Governo è in grado di dotarsi è talmente poco credibile da essere in grado soltanto di alimentare la nascita e la proliferazione di sigle a difesa del Sud. Sud. Il Parlamento, mai come oggi, e mai come in questa legislatura, è stato umiliato e mortificato da una valanga di decreti-legge e di voti di fiducia, da mercati di parlamentari e adesso da documenti sostanzialmente e politicamente superati.

Berlusconi ha chiesto la fiducia alle Camere, con un programma di fine legislatura che è la fotocopia esatta di quello presentato agli italiani già nel 1994 e riproposto poi nel 2001 e nel 2008. in quest'ultima occasione di pochi giorni fa, Berlusconi ha ripetuto di voler completare la riforma liberale che aveva annunciato con la sua discesa in campo e che assicura - ci ha detto - il principio fondamentale del «tutto è consentito, tranne ciò che è vietato».

Ne sanno qualcosa i Comuni, con l'ICI; i contribuenti, con l'Alitalia; le imprese, con l'IRAP; le famiglie, con il *bonus* prima e il quoziente familiare dopo; la Campania, con i rifiuti; L'Aquila, con la ricostruzione. Sapete benissimo che state prendendo in giro gli italiani, perché il percorso di riduzione del debito pubblico delineato dal nuovo Patto di stabilità implica dinamiche di entrata e di spesa credibili solo se l'economia riprenderà a crescere. Sapete altrettanto bene che sono del tutto evanescenti le promesse di una riduzione graduale delle tasse su famiglie e imprese perché, se per le prime il quoziente familiare è soltanto un oggetto misterioso, per le seconde la riduzione dell'IRAP è di fatto un onere a totale carico delle Regioni, che non si capisce come potranno finanziarlo, dopo i tagli

Viviamo in una realtà che è fatta di bassa crescita, di disoccupazione giovanile, di una disoccupazione arrivata nel Mezzogiorno quasi al 50 per cento, di una situazione esplosiva di emergenza per 500.000 famiglie che hanno perso il posto di lavoro e per e per altre 300.000 che lo perderanno, quando sarà finita la cassa integrazione o il periodo di mobilità. Viviamo in una realtà di imprese che chiudono e di un'amministrazione pubblica in un progressivo degrado e decadimento, perché sempre più succube di scelte sbagliate.

il dato Eurostat, in base al quale il reddito *pro capite* degli italiani, che superava di 17 punti il reddito medio europeo, oggi invece è inferiore di quindi, che abbiamo reagito bene alla crisi economica e non è vero che lo abbiamo fatto meglio di altri. Il Paese ci chiedeva più giustizia sociale e più uguaglianza; ci chiedeva di detassare i redditi da lavoro per tassare patrimoni e rendite. Voi non avete fatto nulla di tutto questo; anzi, avete fatto peggio: avete votato lo scudo fiscale per gli evasori, gli elusori e i bancarottieri. Siete gli unici a non capire perché un Governo che voleva spacciare una politica del fare viene accusato dal mondo delle imprese di non riuscire a fare le riforme; siete gli unici a non capire che persino la Chiesa, con il cardinale Bagnasco, ha speso parole di preoccupazione, angustiata, al pari degli italiani, per il degrado della politica. Per non parlare poi del piano Marshall per il Sud. Nel luglio 2009 era stato annunciato un piano di infrastrutture e investimenti per il Sud, ma oggi state ancora

a questa farsa, al teatrino di votare un documento già politicamente e sostanzialmente superato. Non parteciperemo al voto perché la differenza tra noi e voi è che noi pensiamo che il danno maggiore che si possa fare al nostro Paese non è il deficit del 5,3 per cento del bilancio, 5,3 per cento del bilancio, ma il deficit di senso dello Stato, di rispetto per le istituzioni, di attenzione per gli interessi generali, di preoccupazione per le parti più deboli. E questo è l'unico deficit è l'unico deficit che può essere sanato con un semplice taglio: il taglio di questo Governo. Per tale ragione non parteciperemo al voto.

perché non farò l'intervento che mi ero ripromessa di svolgere e rispetto al quale avevo cercato di studiare questa Decisione nei suoi contenuti.

e di un eventuale impegno per tutti i settori dello sviluppo, non certamente dell'assistenza, o di quelli che sarebbero potuti essere gli interventi del Governo prima ancora dell'attuazione del federalismo fiscale. però è accaduto qualcosa di molto più importante in quest'Aula, che ha avuto una valenza politica ancora più forte dei contenuti della Decisione stessa.

pur nella disattenzione totale del Governo e ha cercato di convergere, con molta buona volontà, rispetto ad indicazioni ed indirizzi. Ci

la responsabilità di portare avanti gli impegni enunciati nelle diverse sedi. L'aver affermato che ci si vuole impegnare prioritariamente per il Mezzogiorno sul sul tema delle infrastrutture e della fiscalità di vantaggio è indubbiamente un fatto che ha una sua rilevanza di principio, ma che deve essere tradotto in atti. L'andamento di questa seduta L'andamento di questa seduta evidenzia, da un lato, l'attivismo dei senatori, che hanno cercato di convergere su una questione di principio, su un fatto di indirizzo e, dall'altro, il silenzio totale

oppure che ci desse delle indicazioni anche temporali abbastanza cogenti, spiegandoci quando e come avremmo potuto vedere riflesso nella realtà

circa la guerra valutaria tra Stati Uniti d'America e Cina; però è altrettanto evidente che ciò peggiora le prospettive.

già si accennano rischi di impennata dell'inflazione e, quindi, dei tassi di interesse, circostanza che con il nostro debito pubblico ha i risvolti che tutti conosciamo. Addirittura è in corso un dibattito in America sulla ripresa di posizioni protezionistiche.

supereranno il rapporto del 100 per cento debito-PIL. Significa che tutto l'Occidente in blocco produce più debito che ricchezza, più debito che lavoro: uno squilibrio che ovviamente non può durare a lungo e che necessita di essere aggiustato. Sicuramente nel lungo periodo si procederà all'aggiustamento, ma - come si suole dire - nel lungo periodo saremo tutti morti.

di tutti i Paesi del Mediterraneo, l'unico che non è stato declassato è il nostro. La stessa Irlanda è stata declassata. Quindi, i famosi PIGS, (maiali) sono stati tutti penalizzati, tranne noi. Che cosa significa questo? Significa che è il mercato a decidere se i parametri di finanza pubblica di un Paese sono buoni o meno. In una situazione di confusione, come quella che stiamo vivendo oggi, non basta più l'antico principio

la prima opportunità, abbiamo una spesa pubblica enorme, ben superiore al 50 per cento del PIL: questo significa che abbiamo enormi margini di miglioramento. Abbiamo un enorme debito pubblico e, quindi, rispetto ad altri, abbiamo - per assurdo - un margine di miglioramento. Abbiamo un patrimonio sicuramente notevole. Quindi, è evidente che per noi il problema non è il settore privato. Abbiamo un problema nel settore pubblico. Il nostro problema è l'eccesso di intermediazione del pubblico. Come disse Reagan, per troppo tempo abbiamo pensato che lo Stato potesse risolvere i problemi. Oggi ci accorgiamo che il problema è lo Stato. Allora come uscirne? Tanti colleghi di maggioranza ed opposizione hanno citato il *report* annuale del World Economic Forum. Il principale fattore di non competitività delle nostre aziende è dato non dalle tasse - come potrebbe pensare chiunque - ma proprio dal peso e dall'inefficienza della burocrazia. Per noi, quindi, la strada è segnata. Il problema è Per la Lega Nord è chiaro che tagliare la spesa non è - come abbiamo sentito più volte nel corso di questo dibattito - un problema, ma un'opportunità. Tagliare la spesa produce ricchezza, e non solo nel medio e nel lungo termine: produce ricchezza anche nel breve termine, nell'immediato. È evidente a tutti che, in Italia, lasciare i quattrini in mano a famiglie ed imprese è meglio che darli ad una pubblica amministrazione spesso inefficiente. Visto che a parole siamo tutti d'accordo sul taglio della spesa pubblica, andiamo a vedere che cosa è stato fatto e ragioniamo in prospettiva su cosa si può fare ancora e in modo migliore con il secondo documento, quello delle riforme. Tutti conosciamo le principali voci di spesa pubblica, che sono pubblica

La vostra Puglia, gestita da Vendola, su questo tema non solo è in difficoltà, ma addirittura mette in discussione il sistema. Vorrei capire quale sia la posizione

al cosiddetto secondo documento che ci impone l'Europa, al programma di riforme, al modo in cui possiamo dare maggiore competitività al nostro sistema. Citiamo qualche esempio, anche prendendo spunto dalle considerazioni svolte

Per noi è assolutamente evidente che in particolare sul tema delle liberalizzazioni bisogna essere chiari. Abbiamo avviato la riforma dell'acqua, consentendo ai privati di gestire il servizio.

credo che, alla luce della discussione odierna e dei molti interventi svolti, emerga con tutta evidenza il fatto che non possiamo contribuire al voto su questo testo, peraltro modificato come avevamo ipotizzato dall'emendamento concordato con il Governo. Infatti, questo voto radica l'illegittimità del disegno di legge di stabilità il Senato della Repubblica. Ad umiliarlo contribuisce il silenzio del Governo, a mio avviso del tutto insensato, ma prima ancora l'atteggiamento pilatesco della Presidenza del Senato, perché non è l'opposizione, non è il nostro Gruppo... Credo che la valutazione che ne fanno sia un'altra, Presidente. Come dicevo, non è l'opposizione, e non è il nostro Gruppo, a non essere stata garantita: non è stato garantito il Senato, il suo ruolo, la sua autonomia, le sue attribuzioni e la sua stessa autorevolezza. Ci dispiace per il collega Viespoli, che credevamo conquistato alle ragioni della democrazia parlamentare, che vediamo arreso di fronte a una convenienza che, conoscendo la volatilità degli impegni assunti dal presidente Berlusconi, gli si svelerà presto del tutto effimera. Sono queste le ragioni essenziali, corredate dalle molte con le quali oggi ci siamo espressi in quest'Aula, per le quali non parteciperemo al voto e per le quali il mio Gruppo lascerà l'Aula del Senato.

Colleghi, per cortesia, consentite al presidente Azzollini di svolgere la sua dichiarazione di voto.

avanzate questo pomeriggio cercano di mettere in ombra, ma a mio avviso non ci riescono, alcune questioni fondamentali poste

è lì che si manifesta l'indirizzo del Parlamento al Governo. Per quel che riguarda le

approvata una risoluzione pienamente idonea allo scopo per la quale è prevista. Di certo, come ho sottolineato, è meglio che tale proposta di risoluzione sia approvata prima della proposizione della legge

che tutti gli elementi fondamentali sono perfettamente inclusi nella risoluzione e ci portano ad una decisione sostanziale. Questo mi pare di poter riaffermare. Invece alcune questioni di fondo vanno poste. che questa risoluzione impegna il Governo ad una manovra di finanza pubblica particolarmente incisiva; che in questa risoluzione per la prima volta i parametri che vengono presi in considerazione e fissati sono molto più penetranti che nel passato; che questa risoluzione costituisce un ponte tra la sessione di bilancio, nazionale per così dire, e la nuova sessione di bilancio europea che partirà dal 2011. Questo è il senso profondo di ciò che stiamo approvando questa sera. È qui che l'autorità del Parlamento si sta manifestando; è in questa nuova presa di coscienza del rapporto tra la Decisione di finanza pubblica nazionale e quella europea che si sostanzia l'atto fondamentale che questa sera andiamo ad approvare,

che prevederà, a partire dal prossimo anno, nuovi tempi, nuove procedure, insomma un miglioramento complessivo della trasparenza della sessione di bilancio; però, anche un impegno molto più importante per il rispetto dei saldi. Questa Decisione di finanza pubblica, peraltro, viene dopo, e certifica, due significativi successi del Governo. Il primo è quello della gestione e conduzione della più grave crisi finanziaria che si ricordi a memoria d'uomo,

nella storia dell'Unione europea di alcuni parametri che vedono l'Italia al vertice o comunque alle primissime posizioni tra le Nazioni europee, e questo significherà che potremo guardare con più serenità alle ipotesi di crescita, perché meno stringente sarà il vincolo di bilancio che verrà non soltanto dai parametri di Maastricht esistenti ma da quelli nuovi che il nostro Governo sta introducendo all'interno dell'Unione europea. Queste sono le questioni sulle quali penso che dobbiamo profondamente riflettere e che inducono il mio Gruppo a votare in maniera convinta a favore della Decisione di finanza pubblica. Ogni ritardo, ogni indecisione sarebbe suonata come irresponsabile, non soltanto nei confronti della Nazione, ma anche dell'Unione europea.

l'Italia contribuirà in maniera fondativa alla sessione di bilancio europea, che i parametri che connotano positivamente la finanza pubblica italiana saranno presi in considerazione e che a partire da questo il Governo si porrà gli obiettivi di crescita che che soli possono garantire e migliorare la coesione sociale del Paese. Non mi soffermerò su tutte le questioni che poi vengono nella narrativa della risoluzione

sono affrontabili soltanto se la nostra economia e la nostra finanza pubblica non cedono di fronte ad una crisi che certo si sta superando, ma che necessita ancora di un'attenzione precisa come quella che il Governo vi sta ponendo in questo momento. Per questo, signora Presidente, colleghi, ci accingiamo a votare con serenità la risoluzione di maggioranza, così come integrata, perché ha specificato meglio le questioni del Mezzogiorno e affrontiamo i cinque punti posti dal presidente del Consiglio Berlusconi innanzi al Parlamento con grande serenità. È il momento della prospettiva, e io credo che questa maggioranza sia l'unica in grado di contribuire ad una prospettiva positiva dell'Italia nell'Unione europea.

Tutti i punti che sono reiterati per il terzo anno consecutivo, anche se di nuova misura si tratta, non si sono mai tradotti in politiche di riforma. La crescita viene ulteriormente, ancora una volta, presentata ma, nei fatti, non c'è. Basterebbe andare a vedere il presunto incremento del nostro commercio internazionale, per poi andare a scoprire che a questo non corrisponde, per esempio, nessun tipo di trattamento di favore che l'Italia avrebbe potuto guadagnare grazie alle frequentazioni del Presidente del Consiglio per quanto riguarda l'approvvigionamento di gas e di petrolio avendo oramai sviluppato un'amicizia fraterna con Putin e con Gheddafi. Per questo motivo, il nostro voto

prevede che il Presidente della Repubblica autorizzi la presentazione dei disegni di legge di iniziativa del Governo alle Camere: e di questo si è trattato. Quindi, forse involontariamente, tutte le censure rivolte, per me ingiustamente,

Signor Ministro, in realtà sarebbe bene tenere fuori - credo - il Presidente della Repubblica da questo dibattito. *(Commenti dai il nostro rispetto è totale per tutti, anche per i Vice Presidenti, perché, come ha detto oggi il senatore Nania, voi presiedete un'Assemblea che può assumere tutte le determinazioni. Voglio associarmi alle parole del ministro Calderoli e sottolineare il senso di responsabilità dei Gruppi di maggioranza, perché è noto che i disegni di legge del Governo debbano seguire una certa procedura. A maggior ragione immagino l'attenzione su un disegno di legge così importante come la legge finanziaria, oggi denominata legge di stabilità. Ed abbiamo voluto evitare, noi, di tirare in ballo una polemica sulle massime istituzioni della Repubblica, che rispettiamo in maniera totale, a differenza evidentemente di altri in quest'Aula del Senato. Voglio anche aggiungere che ringrazio il Governo, perché molti hanno parlato oggi ma non hanno letto i giornali. È vero, sono importanti questi atti parlamentari preliminari alla finanziaria, o meglio, alla legge di stabilità.

quella riunione. Oggi «la Repubblica» - cito il giornale più lontano dalle nostre posizioni, di quelle dei nostri banchi - titola: «Nuovo Patto di stabilità: l'Italia la spunta sul debito», perché il ministro Tremonti, il Governo Berlusconi hanno ottenuto in Europa che accanto ai parametri del debito pubblico, assai gravosi per le ragioni storiche, si tenesse conto, al fine della valutazione delle Nazioni, del risparmio complessivo. E l'Italia è un Paese di risparmiatori. Il principio sostenuto dal nostro Governo è stato accolto in Europa. Queste sono le cose che contano, cari colleghi!

tutta l'indignazione possibile per le parole che ha appena reso il ministro Calderoli. Mi trovo in Aula soltanto per restare vicino alla collega Granaiola che sta per intervenire. Il ministro Calderoli si è

Il Governo è stato più volte invitato ad intervenire per far conoscere la propria opinione. Il ministro Calderoli, insieme ai suoi colleghi e Sottosegretari, si è guardato bene dal prendere la parola e poi,

di aver tirato in ballo il Presidente della Repubblica quando è noto il rispetto che noi abbiamo per il Presidente della Repubblica. È stato il ministro Calderoli, per ragioni strumentali, ad aver tirato in ballo una figura così alta, per cui, se c'è una persona che deve essere richiamata, è il ministro Calderoli, non chi rifiuta di essere tacciato come persona o forza politica che attacca il Presidente della Repubblica. In ogni caso, il *vulnus* c'è stato, lo strappo da parte del Governo nei confronti del Parlamento si è verificato ed io sono convinto che chi ha avuto modo di seguire questo dibattito avrà potuto verificare l'arroganza, la supponenza e il dileggio con i quali il Governo ha trattato non solo le opposizioni ma tutto il Senato.

Signora Presidente, chiedo nuovamente di intervenire sul caso di Daniele Franceschi, il ragazzo di Viareggio morto nel carcere di Grasse, dove era detenuto dal febbraio scorso in attesa di essere processato con l'accusa di aver usato al casinò una carta di credito falsa. Dopo quel decesso, causato con molta probabilità da una scarsa considerazione delle condizioni del ragazzo, che aveva supplicato per iscritto, addirittura in francese, di essere visitato per i forti dolori al petto e alla spalla, è stato un susseguirsi di eventi a dir poco sconcertanti: dopo l'autopsia, addirittura ci si dimentica di mettere il corpo in frigorifero. Su quel corpo, al quale sono state effettuate molteplici amputazioni, compresi gli occhi, in stato avanzato di decomposizione, come e con quali risultati potrà essere eseguita quella nuova autopsia ottenuta con grande fatica dagli avvocati e autorizzata finalmente dalla procura di Lucca? Ho posto dei quesiti al ministro Frattini tramite il presidente Schifani, che ringrazio. Ho chiesto alla Commissione d'inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale, ove possibile, di intervenire per fare chiarezza sulla vicenda. Mi auguro che tutto il Senato, al di là degli schieramenti, faccia propria l'esigenza di fare il prima possibile luce sull'accaduto, senza attendere che sia solo un intervento di Carla Bruni - peraltro auspicabile e gradito - a smuovere le autorità giudiziarie francesi. Occorre chiedere che sia fatta giustizia: eventi terribili come quello di Daniele Franceschi non devono mai più accadere. Domani vedrò il ministro Frattini: vorrei aggiungere alla mia determinazione e a quella del console generale di Nizza Agostino Chiesa Alciator quella di tutti i colleghi. È il minimo che possiamo fare per una madre che, per aver protestato, sia pure violentemente, davanti al carcere per non poter dare l'ultimo saluto al figlio, è stata arrestata e buttata a terra, con conseguente frattura delle costole. È il minimo che possiamo fare, per la dignità di ogni essere umano, anche se ha sbagliato, anche se è detenuto.

a grappolo: esso è stato comunicato alla Presidenza del Senato il 3 agosto 2010, ha come primi firmatari la senatrice Pinotti e il senatore Casson concerne in particolare la ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla messa al bando delle munizioni a grappolo aperta alla firma a Oslo il 3 dicembre 2008.

dei sindacati autonomi di Polizia penitenziaria, il SAPPE, contro l'immobilismo asfissiante e l'apatia dei vertici del DAP rispetto ai problemi quotidiani della Polizia penitenziaria e contro la colpevole indifferenza di questo Governo ai gravissimi problemi penitenziari. Gli appartenenti al SAPPE, ma anche, lo ripeto, tutti i lavoratori della Polizia penitenziaria, rivendicano le più volte annunciate assunzioni che questo Governo promette periodicamente attraverso il ministro Alfano, che ha parlato di assunzioni di 2.000 agenti della Polizia penitenziaria, nonché di provvedimenti concreti per risolvere l'emergenza delle carceri. I lavoratori chiedono il pagamento del lavoro straordinario già espletato e svolto obbligatoriamente, il pagamento delle competenze per i servizi di missione dei nuclei traduzioni e i piantonamenti, e le risorse necessarie all'ammodernamento degli automezzi e per il vestiario. Oggi è stata approvata la Decisione di finanza pubblica, che tutto fa, meno che tutelare i lavoratori che ci hanno consegnato questa maglietta per il Senato.

allontanato o addirittura disilluso con le parole del ministro Alfano. Era un dovere rappresentare questa protesta della Polizia penitenziaria, perché, oltre alla lotta che noi tutti portiamo avanti a tutela della persona del detenuto, dobbiamo anche rivolgere un'attenzione particolare a chi tutti i giorni vive insieme al detenuto: e questa persona è nella figura della Polizia penitenziaria. **Per

ossia da ben 110 giorni, dopo l'ingloriosa uscita dell'ex presidente Cardia, destinato dal Governo ad altri ben retribuiti incarichi. Nel sollecitare ancora una volta a provvedere alla nomina di un presidente e di un commissario (posto che il presidente vicario Conti non sembra adatto a reggere il timone di una Commissione importante, soprattutto in una fase di crisi come questa, con equità ed equilibrio, dati i suoi trascorsi in una grande banca),

che riguarda "parentopoli" alla CONSOB, ossia il sistema di assumere persone per chiamata diretta senza concorsi di evidenza pubblica e che poi, tramite concorsi interni pilotati, come

2010, che riguardava le retribuzioni all'interno della Banca d'Italia, tenendo conto che proprio qualche giorno fa abbiamo letto alcune veline sui giornali riportate in maniera acritica da giornalisti (probabilmente erano funzionali), su un taglio del 10 per cento degli stipendi del direttorio

signora Presidente, il Governo rispondesse a questa interrogazione. Vorremmo sapere quanto guadagnano perché, tra l'altro, ci sono ispettori che fanno le ispezioni e che, magari, fanno assumere anche le amanti.

antecedenti la presentazione delle liste elettorali, in particolare nella Regione Lombardia. Lunedì 1° marzo 2010, a seguito delle verifiche effettuate in sede di visione degli atti, Lorenzo Lipparini - delegato della lista Bonino-Pannella per la Lombardia - depositava presso il medesimo Ufficio elettorale centrale della Lombardia un esposto nel quale veniva segnalata una serie di ritenute irregolarità nelle sottoscrizioni apposte dai presentatori dei "listini" regionali. Nell'esposto venivano segnalate in particolare: la mancanza dei timbri degli autenticatori, la data e il luogo di autenticazione delle firme, la presenza di certificati elettorali richiesti e stampati in un momento antecedente rispetto a quello in cui ciascun presentatore risultava aver apposto la propria sottoscrizione (circostanza evincibile dalla data di autenticazione delle sottoscrizioni stesse). Lo stesso giorno 1° marzo 2010, Marco Cappato - candidato per la lista Bonino-Pannella alla presidenza della Regione Lombardia - e Lorenzo Lipparini depositavano un esposto-denuncia presso la procura della Repubblica presso il tribunale di Milano, al fine di sollecitare delle indagini in particolar in particolar modo in ordine a possibili reati di falso di cui risultavano alcune evidenze sul listino di Formigoni, òe cui firme, anche in base a dichiarazioni pubbliche provenienti da soggetti di quello schieramento politico, oltre che a varia documentazione, pure resa pubblica, sarebbero state in gran parte autenticate in date anteriori al 24 febbraio, giorno in cui, sempre sulla base di notizie di pubblica notorietà e a interviste rilasciate dallo stesso Formigoni, sarebbe stata definita la lista dei candidati a sostegno di Formigoni. Inoltre, gli esponenti Marco Cappato e Lorenzo Lipparini segnalavano anche una grande somiglianza di calligrafia in molte delle sottoscrizioni apposte sui moduli, chiedendo espressamente il sequestro degli stessi. Contestualmente veniva presentato un esposto avente ad oggetto le sottoscrizioni apposte dai presentatori del listino del candidato Penati. Questa mi pare una questione di grandissima attualità, non soltanto perché sono state presentate le perizie calligrafiche, ma anche perché il quotidiano «la Repubblica», nella sua edizione regionale di Milano, ha condotto delle indagini indipendenti da cui stanno emergendo ulteriori elementi che sicuramente dovranno essere acquisiti dalla magistratura.